l'impressione che il sistema non funzioni, ma il sistema tornerà a funzionare quando dichiarerò aperta - cosa che sto facendo - la verifica del numero legale.

Si presume che quando si viene in Aula si debba votare; per poterlo fare, bisogna avere la tessera.

Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Onorevoli colleghi, grazie per l'attenzione che porrete alla questione e per gli spunti di riflessione che vorrete apportare alla nostra discussione. Grazie all'onorevole Fassina per la sua presenza sui banchi ci troviamo oggi a discutere una questione per noi molto importante sotto l'aspetto politico, economico e di politica industriale. Tale questione riguarda, appunto, le modalità secondo le quali vengono selezionati, valutati e quindi scelti i dirigenti delle società a partecipazione statale, tra cui troviamo, per le questioni più urgenti, quella del rinnovo del consiglio di amministrazione di Finmeccanica, ma anche la questione più imbarazzante, cioè il caso di caso di ENI. Quello della poca trasparenza delle procedure di nomina dei consigli delle società a partecipazione statale è un problema che non può più essere rinviato, perché riteniamo sia giunto il momento di attribuire ai cittadini un reale potere di intervento nell'individuazione degli organi di governo di enti di primaria importanza. Vorrei sottolineare subito che questa nostra iniziativa non è passata inosservata e che nelle scorse settimane si è assistito ad un fermento di notizie e fatti al riguardo. Non è passata inosservata al mondo industriale, perché all'atto della pubblicazione della nostra mozione abbiamo ricevuto sostegno e soprattutto informazioni preziose da parte di un gruppo di lavoratori di una azienda collegata a Finmeccanica, che si sono autodefiniti «dipendenti puliti». Abbiamo ricevuto inoltre segnalazioni e commenti da parte di dipendenti di ENAV e Selex e anche su Fincantieri. Non è passata inosservata infine al nuovo Governo, il quale, come riportato dal «Il Sole 24 ORE», in data 29 aprile, ha chiesto il rinvio della nomina di alcuni membri del consiglio di amministrazione di Finmeccanica, a garanzia di trasparenza di questa fase, per permettere al Governo stesso di intervenire con sue proposte. Tutto questo, onorevoli colleghi, a testimonianza del grande interesse generale sulla questione. Fino ad arrivare poi ad oggigiorno, in cui sappiamo che il consiglio di amministrazione di Finmeccanica ha prorogato la nomina al prossimo luglio e che abbiamo tre mozioni all'ordine del giorno sulle quali discutere.

Vorrei parlare innanzitutto del dramma di Finmeccanica, che non è dato solo dalle inchieste giudiziarie, che faranno il loro giusto corso, ma anche dalla paralisi che esse provocano nel più delicato e strategico gruppo industriale italiano. Il dramma non è solo avere un ex presidente e amministratore delegato, tal Giuseppe Orsi, indagato per corruzione internazionale, riciclaggio e illecito finanziamento ai partiti, ma è anche avere un Governo paralizzato dall'imbarazzo e incapace di prendere una decisione. Eppure stiamo parlando di 70.000 posti di lavoro, legati alla produzione di aerei, di elettronica, di elettronica di sistema, di centrali elettriche e treni. Ecco allora che oggi in quest'Aula abbiamo noi tutti una grande occasione per dimostrare che la politica è ancora in grado di tutelare gli interessi nazionali e dei cittadini interessi che sono ascrivibili nella categoria dei beni comuni, non già essenziali nella loro accezione generica, ma fondanti e basilari, come la nostra Costituzione ci ricorda nel suo grido di apertura. Ed uso la parola grido non a caso, signori, perché un principio disatteso non può che essere e trasformarsi in un grido di riscatto. È possibile, a ragione, parlare di bene comune, perché con partecipazioni statali raccontiamo una storia tutta italiana che nasce nei primi del Novecento, si sviluppa e consolida con il *boom* economico

(1953). Noi oggi siamo chiamati ad un grande atto di responsabilità verso questo patrimonio comune che sono le partecipazioni statali. Ma non solo. Possiamo essere anche di esempio e guida per le migliaia di partecipazioni degli enti locali. Permettetemi allora di entrare più in dettaglio, ricordando che Finmeccanica, prima delle 31 società a partecipazione statale a rinnovare il suo consiglio di amministrazione, è una delle realtà industriali più importanti del Paese, presente in settori strategici, capace di operare e competere in ambiti internazionali. La *holding* è attiva nei settori dell'aeronautica, dell'elicotteristica, dell'elettronica applicata alle tecnologie satellitari e alle telecomunicazioni, dei sistemi di controllo delle reti di trasporto ed energia, negli apparati per la produzione di energia elettrica. Ma soprattutto, Finmeccanica ha una *leadership* tecnologica riconosciuta e consolidata in progettazione, sviluppo e produzione di sistemi missilistici, siluri, artiglieria navale e veicoli corazzati. Questi aspetti, in particolare l'ultimo, determinano una condizione di necessità di massima trasparenza nelle funzioni di amministrazione di questa società. La stessa condizione di necessità la troviamo anche in ENI. L'Ente nazionale idrocarburi, creato da Enrico Mattei, è la più grande e strategica impresa italiana, con un fatturato annuo di 100 miliardi di euro, 79.000 dipendenti, operante in 85 Paesi principalmente nel settore dell'energia.

è Paolo Scaroni. Il Governo ha promesso nuovi criteri di nomina per gli amministratori delle società pubbliche per introdurre trasparenza e merito ed evitare che i pilastri di quel che resta dell'industria italiana (ENI, ENEL, Finmeccanica) vengano consegnati nelle mani di incapaci con amici influenti. Questa è un'ottima notizia; tuttavia, la cronaca recente ha dimostrato che la politica è stata completamente incapace di prendere decisioni operative così importanti. Infatti, Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI, è indagato per corruzione internazionale, ma nessuno ne ha chiesto le dimissioni. Chi ha buona memoria ricorderà anche che la cosiddetta Prima Repubblica si sbriciolò a causa delle tangenti Enimont. Nel 1992, proprio durante il periodo di Mani pulite, Scaroni finì in manette, e nel 1996 patteggiò una pena ad un anno e quattro mesi di carcere per tangenti di svariate centinaia di milioni di lire, versate al Partito Socialista Italiano per ottenere l'assegnazione di appalti all'ENEL, azienda allora guidata dallo stesso *manager*. Da ultimo, nell'assemblea dello scorso maggio di ENI, la Fondazione culturale responsabilità etica (Banca etica), uno degli azionisti di ENI, ha portato all'attenzione la sospetta corruzione in Algeria che ha coinvolto ENI e la controllata Saipem all'inizio dell'anno. In base alle ricostruzioni della procura di Milano, il gruppo ENI avrebbe pagato circa 200 milioni di euro a "faccendieri ed esponenti del Governo algerino" per assicurarsi commesse (tra cui la costruzione di un gasdotto nel Nord Est del Paese) dal 2006 al 2010. Parte del denaro sarebbe poi rientrata sui conti di alcuni *manager* italiani Oltre al profilo morale è bene sottolineare anche alcune note sotto il profilo tecnico della questione ENI. Ad esempio, possiamo segnalare scelte manageriali discutibili, quali, ad esempio, la stipula di contratti poco lungimiranti del tipo *take or pay*, senza previsioni reali di distribuzione, che fanno pensare a scelte poco oculate dei livelli dirigenziali. Per non parlare poi del fatto che i contratti sono a prezzi vincolati al mercato del petrolio, il che, parlando di gas naturale, sembra quasi un ossimoro. Alla luce degli appelli e delle richieste che provengono da molteplici settori dell'opinione pubblica e della società civile, ma anche al fine di evitare il ripetersi di episodi che hanno visto il coinvolgimento di parte del *management* di Finmeccanica e di ENI in questioni che appaiono senz'altro censurabili sotto il profilo dell'opportunità e in grado di mettere a rischio non soltanto la credibilità dell'intera struttura manageriale ma anche la competitività di alcune delle più importanti aziende italiane, è ancora possibile dare al Paese un importante segnale di discontinuità, mettendo in primo piano l'esigenza di una forte trasparenza nel procedimento di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione di queste, come delle più importanti società italiane. Finmeccanica, ENI e tutte le altre, pena il proprio declino, hanno l'estrema necessità di tutelare l'immagine aziendale, l'onorabilità del marchio e la serietà della struttura industriale e non possono essere guidate in futuro da un *management* che opera in controtendenza rispetto alla corretta gestione aziendale. Chiarita allora la situazione generale, indico le premesse per le richieste di questa mozione. Tali premesse sono circoscrivibili soprattutto in termini di impegno in trasparenza e scelte che conducano a reali, pari opportunità. Impegni però che dobbiamo essere in grado di trasformare in vere opportunità. Per questo,

alla nomina mediante esami trasparenti di candidature ricevute con bando pubblico sempre su sito *web* del Ministero, e previa pubblicazione dei *curricula* ricevuti; a rendere pubblici i *curricula* dei candidati anche agli *stakeholder* principali dell'azienda; a permettere la verifica delle proposte governative di nomina anche al parere delle Commissioni competenti, superando il tentativo di far divenire prassi l'istituzione di Commissioni di saggi in *real time.* in *real time.* Oggi abbiamo quattro punti da discutere insieme, e spero vivamente anche da approvare insieme, in tempi rapidi per dare un grande segnale di innovazione metodologica nel nostro Paese; per dimostrare che, in un'analisi che potremmo definire politico-antropologica, è finalmente chiusa l'era politica pre 5 Stelle, e che arriveremo in questo modo, magari un giorno, ad applicare un principio democratico importante, e per noi fondamentale. Sto parlando del principio secondo il quale una cosa che riguarda tutti, deve essere decisa da tutti. Questo per permettere ora ad alcune delle più importanti aziende italiane di riprendere la loro storia con modalità ispirate a principi di

signor Vice Ministro, la ringrazio per la presenza perché la sua è una presenza qualificata, anche per storia personale e non solo per ruolo; ci intenderemo su alcuni passaggi, che non sono semplicemente quelli esplicitati all'interno del dispositivo ma fanno parte di un ragionamento un po' più ampio. Di fatto,

Nella precedente legislatura - lei forse si ricorderà, avendo seguito, seppure dall'esterno, questi particolari argomenti - si tentò anche di fare una mappatura concreta, e non semplicemente riferita alle 31 partecipazioni dirette che il Tesoro ha all'interno di società, di una serie di condizioni di presenze all'interno di una grande, enorme forse, serie di controllate e partecipate. Tornando indietro con la memoria, e anticipando che questa società non c'è più, qualche anno fa mi capitò di vedere una società dello Stato, che tra l'altro operava in una particolare area d'Italia - mi riferisco

al livello di *management,* delle società che sono controllate. Lei me lo insegna, e sa che, per ora, per norma e anche per consuetudine, lo stesso Tesoro all'interno dei consigli di amministrazione

modo, molti dipendenti, funzionari e dirigenti del pubblico sono, per esempio, presidenti dei comitati compensi; quindi, sarebbe interessante analizzare anche questo profilo, cioè il fatto che non prendano compensi come consiglieri di amministrazione ma li prendano invece come presidenti

lavoro comunque propedeutico alla loro azienda, si siedono nell'anticamera di un Ministro, oppure vanno a fare il loro lavoro di rapporto o contatto, magari con qualche *authority*. Signor Vice Ministro, lei sa come me che noi quelli non li conosciamo. Gli amici e colleghi del Movimento 5 Stelle hanno proposto la mozione indicando nomi di aziende e di persone che normalmente si leggono nelle prime pagine dei giornali

C'è un ultimo passaggio, Vice Ministro, che riguarda i compensi. Voi abbiamo già stato posto un limite ai compensi: ci riproviamo; sappiamo che non è mai stato facile e che, anzi, ci sono state proposizioni per cui determinate situazioni non si possono toccare, ma

mozione di trasparenza. Pensiamo che possa essere apprezzabile, lo diciamo anche avendo vissuto vicende dalle quali ci siamo dissociati, ma che - a differenza di altri - non facciamo finta di non conoscere.

di grande impatto sull'opinione pubblica, perché riguarda la *governance* di società partecipate dallo Stato, in questo caso attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze.

e del Governo e la necessaria richiesta, che sale impetuosa dall'opinione pubblica, di gestire anche passaggi così delicati e importanti all'insegna della trasparenza e del rispetto quanto più puntuale possibile dei profili di professionalità. In questi ultimi anni il processo di dismissione delle partecipazioni pubbliche al complesso delle società che hanno rilevanza nel tessuto economico, produttivo e industriale del Paese ha portato a ridurre fortemente la presenza dello Stato, pur conservando questo poteri di indirizzo e di nomina degli amministratori. Il tema si pone dunque in termini di attualità, rispetto alla necessaria assunzione di responsabilità che credo tocchi alla politica e alle sue istituzioni, a cominciare dal Parlamento, che può e deve offrire al Governo e ai Ministeri direttamente coinvolti degli indirizzi puntuali, rispetto ai criteri e alle procedure che vanno e che possono essere seguiti. parlando di società importanti, su cui negli ultimi anni è intervenuta una mole di attività legislative, che ne ha fortemente trasformato le caratteristiche giuridiche, la *governance* e l'organizzazione interna. società su cui hanno impattato norme, che riguardano più complessivamente il perimetro pubblico, a cominciare dagli interventi della cosiddetta *spending review*, che hanno votato e ispirato alcune scelte ai principi di efficienza e di efficacia, da raggiungere anche con il contenimento

nel misurare quella discrezionalità che le istituzioni, e con esse la politica, possono e devono rivendicare, però dentro un quadro di indirizzi che oggi, con questa discussione,

per la composizione degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale che oltre a garantire un'adeguata rappresentanza di genere voglio ricordarlo - in linea con la più avanzata e stringente normativa adottata dal nostro Paese negli ultimi tempi, siano altresì assicurati, soprattutto, i requisiti di trasparenza e di certezza nei criteri e nelle procedure di nomina e decadenza dei componenti degli stessi organi amministrativi delle società di cui stiamo parlando. In particolare, l'attuale sistema prevede già il rispetto dei requisiti di onorabilità, accanto ai quali è necessario introdurre, a nostro parere, ulteriori requisiti e limitazioni alla nomina dei componenti dei consigli di amministrazione, con riferimento in particolare ai requisiti soggettivi, nel caso ad esempio di

cariche negli enti locali, nelle Regioni, nei consigli di amministrazione, nello stesso Parlamento italiano o in quello europeo.

congruo di incarichi in analoga responsabilità, esperienza nel settore industriale di riferimento, autorevolezza adeguata all'incarico, verificabilità della reputazione e della riconoscibilità sui mercati di riferimento, assenza di conflitti d'interesse o cumulo di cariche in società concorrenti. La mozione indica espressamente l'attivazione, peraltro, di una valutazione comparativa dei requisiti professionali richiesti. Questo mi pare un elemento di grande innovazione su un tema così delicato

vi sono parti assolutamente condivisibili e altre che lo sono meno, ma voglio dire ai colleghi della Lega e del Movimento 5 Stelle che la nostra mozione su questo punto in particolare, se mi è concesso,

chiediamo al Governo di attivare procedure di valutazione comparata dei *curricula* o comunque di coloro i quali manifesteranno interesse e disponibilità a concorrere ad occupare posti così delicati di comando comando nelle aziende partecipate pubbliche, che sono, ripeto, di eccellenza e particolarmente significative. Per quanto attiene poi, nello specifico, alle procedure di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società, riteniamo necessario che vengano rispettati determinati requisiti di trasparenza e pubblicità; anche questo è un tema che condividiamo con le altre mozioni, ma ci permettiamo di dire qualcosa in più e di individuare una procedura, attraverso la pubblicazione sui siti dei Ministeri interessati e delle società controllanti e controllate. Insomma, si tratta di un'assunzione di responsabilità piena ed una sfida vera ad accogliere il tema della trasparenza e della verificabilità dei processi decisionali che presiedono a scelte così significative. Ritengo inoltre importante, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previsti per le nomine, che le stesse siano sottoposte ad un monitoraggio, attraverso lo svolgimento, da parte del Dipartimento del Tesoro, di una sorta di istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale sulle candidature e su altre disponibilità, a seguito della quale le nomine stesse potranno essere sottoposte a loro volta ad un comitato di garanzia che abbia il carattere della stabilità e dell'imparzialità e sia competente nelle materie di cui qui parliamo.

Auspichiamo che il Governo voglia accogliere gli indirizzi suggeriti in questa nostra mozione e che gli impegni che abbiamo qui esplicitato con quest'atto possano essere fatti propri anche quest'atto possano essere fatti propri anche dalle altre pubbliche amministrazioni. Chiediamo conseguentemente al Governo che anche su questo ultimo punto possa esservi un impegno conseguente. Nel contempo,

vincolanti e trasparenti, voglio auspicare davvero che vi sia la più larga coesione è coincidenza di vedute, nonché il più largo consenso da parte dell'intero Senato su questo testo così circostanziato e impegnativo che abbiamo depositato. *(Applausi

ci troviamo di fronte alla cura del sintomo e non all'eradicazione della causa del male. I tempi che corrono sono tali sono tali da indurre la politica a dare segnali di trasparenza, di competenza e di moralizzazione. Ben venga tutto questo,

«L'iniziativa economica privata è libera». I Costituenti però non vollero fermarsi a questo primo capoverso che, di per se stesso, ritengo esaustivo, vollero, in quel clima di compromesso tra il più grande partito della sinistra e le forze laiche e democristiane, aggiungere:

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». È da questo secondo capoverso che nasce la triste storia dello Stato imprenditore. Chi ha avuto modo di leggere «Lo Stato onnipotente» di Ludwig von Mises sa bene quanto è costato lo Stato imprenditore. Ancora oggi, nel momento in cui il debito pubblico, che è gran parte figlio di quelle dissennate partecipazioni dello Stato alla libera iniziativa economica, delle sue interferenze, dei monopoli che lo Stato pretende ogni qual volta cerca di fare l'imprenditore, ancorché privo di qualsiasi riferimento alla legge della libera economia e senza alcun criterio di controllo terzo della produttività, del merito, dell'efficienza e dell'economicità, noi siamo qui a legiferare e a normare con delle mozioni le modalità di composizione dei consigli di amministrazione. Siamo qui a somministrare una moralistica aspirina ad un malato grave, che è in gran parte causa di 2.000 miliardi di euro di debito. Ebbene, Luigi Sturzo, nel lontano 1954, ammoniva in questa Aula sulle tre «male bestie» che avrebbero avrebbero affamato e ridotto la democrazia parlamentare italiana: lo statalismo, la partitocrazia e lo spreco del pubblico denaro. denaro. Questi tre elementi sono tutti contenuti, se non incarnati essi stessi, all'interno della gestione dei monopoli o delle partecipazioni dello Stato alla libera iniziativa.

la pianificazione era lo strumento politico portante, che distingueva questo tipo di società e di Stato politico?

Filadelfia si è scelto Parigi con la nostra Costituzione: non abbiamo scelto un cittadino che si serve dello Stato, ma uno Stato opprimente e pervasivo che pretende di fare l'imprenditore, il medico, il pedagogo e ogni altra attività nel campo dell'economia attraverso le partecipazioni statali. Qualunque sia la mozione che andremo ad approvare sappiate, colleghi senatori, che si tratta di un'operazione di mera facciata che corregge i sintomi, ma non cura le cause. È lo statalismo, è la funzione dello Stato nell'impresa il vero nemico della libertà economica. questa dicotomia tra libertà e liberismo fu fonte di dibattito tra Croce ed Einaudi - il barone Compagna forse lo direbbe meglio di me disse a Croce che la prima delle libertà era quella di intraprendere, la libertà di fare; questa non può essere mutuata né condizionata né avvilita né orientata né coordinata da uno Stato che come libera espressione di libere volontà non è nato per fare l'imprenditore se non per fare clientelismo, sperpero del pubblico denaro, occupazione di posti di potere e di sottogoverno da parte delle forze politiche, dilapidando risorse che in mano alla vera iniziativa privata porterebbero ricchezza a questa Nazione. Non mi attarderei, come ha fatto il collega del Movimento 5 Stelle, nell'andare ad evidenziare le ruberie e le distorsioni del sistema. Prima Repubblica è andata a casa per una tangente di 300 miliardi di lire, ma nessuno in questa Nazione ha ancora denunciato e pagato i 2.000 miliardi di lire che lo Stato sperperò vendendo e comprando da Gardini le azioni Enimont, solo perché quest'ultimo voleva rendere la chimica italiana efficiente chiudendo tutte le industrie decotte che servivano da ammortizzatori sociali. sociali. Di che cosa vogliamo allora parlare qui dentro oggi? Vogliamo parlare dell'ILVA, della Telecom, di tutto ciò che con l'Enimont lo Stato ha dismesso e svenduto e che sarebbe pronto a ricomprare qualora questi tipi di ambiti e di interventi dello Stato stesso mettessero in discussione il sottogoverno e il sottopotere che viene dalla partecipazione dello Stato Come si fa, colleghi senatori, a non vedere che la prima e vera causa dello sfascio dei conti dello Stato è lo Stato stesso, la sua pretesa di essere imprenditore, di essere tutto ciò che non doveva essere? Orbene, il Governo delle larghe intese credo abbia un senso se utilizza il vasto consenso parlamentare di cui dispone per eradicare le cause del male, non per fare impacchi o cure palliative ad una Nazione ormai agonizzante.

veramente una diversa attenzione e non solo per le modalità di nomina degli amministratori delle società controllate e partecipate dalla pubblica amministrazione, ma soprattutto per la dimensione molto ampia di questa categoria di soggetti sostanzialmente pubblici, anche se si configurano spesso in forme privatistiche. Non sono sicuro di aver trovato la pagina giusta nel sito del Ministero della funzione pubblica, non so se il Governo aggiorna

legge su tale sito: «Nell'ambito dell'Operazione Trasparenza il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione pubblica pubblica *online* l'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da

parla di 2.365 consorzi, a 4.741 società partecipati dalla pubblica amministrazione e soprattutto di 24.713 rappresentanti, ossia consiglieri di amministrazione a vario titolo impegnati nel governo di questo mostro

dato preoccupa maggiormente in ragione dell'articolazione territoriale delle nostre società partecipate

il numero stragrande dei soggetti di questo tipo è allocato nel Centro-Nord, ricco e potente, cioè quello dell'iniziativa privata

il numero minore lo troviamo nel Lazio, nella Sardegna e nella Sicilia. Sono andato a stamparmi qualche pagina, ma poi ho smesso, perché l'elenco è di 1.295 pagine. Non ho stampato neppure l'elenco di coloro che governano questo mostro, almeno al 2009 (i dati del 2010, infatti, forse non li abbiamo ancora).

significativi emolumenti per governare strutture la cui funzione, consistenza, qualità e utilità è tutta da verificare.

ciò che però non possiamo tollerare è la moltiplicazione dei soggetti pubblici, quelli legittimamente discendenti dal presupposto giuridico del nostro ordinamento: le nostre pubbliche amministrazioni e i nostri enti locali. Stiamo abolendo le Province, perché sono un sovrappiù, ma se abbiamo 25.000 soggetti a forma privatistica che fanno di tutto e di più, che non sono sottoposti ad un controllo serio e che garantiscono nomine di tipo clientelare, allora di che cosa parliamo? *(Applausi una modalità democratica di selezione di un gruppo dirigente che deve governare i problemi di un territorio, gli interessi e le aspirazioni e soddisfare i bisogni di comunità? Signor Presidente, noi siamo interessati, ma - lo dico ai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, ma anche agli agli altri presentatori delle mozioni - non abbiamo presentato mozioni. Condividiamo gran parte delle cose che sono state sollevate, ivi compresa la questione di genere, che andrebbe poi vista nel dettaglio. Magari le funzioni più importanti, nelle società più importanti, non sono affidate alle donne, magari - tra i 25.000 amministratori a vario titolo dispersi in questo ciclopico e numerosissimo in questo ciclopico e numerosissimo sistema di società ci sono anche donne che amministrano (e forse amministrano anche bene nelle realtà dove fanno); a noi, però, interessa di più, che le selezioni avvengano secondo il principio che deve presiedere a tutte le funzioni pubbliche:

alla militanza in un partito, o di un premio - o, meglio, di un'opportunità - di reddito in ragione di qualche favore ottenuto; tanto meno deve essere uno strumento di governo di cosa pubblica a fini direttamente connessi ad una formazione politica, ad un gruppo di interessi o ad una persona fisica. Pensiamo cioè che debba andare avanti un percorso di moralizzazione, senza tentennamento alcuno. Lo dico al Vice Ministro: forse varrebbe la pena capire qual è la consistenza vera di questo sistema e, una volta avuti i dati, fare un dibattito più compiuto su questo argomento (magari su una relazione del Governo).

un numero importante di società di cui il Ministero dell'economia, per conto dello Stato, detiene partecipazioni parziali o totali. In realtà, non si tratta di un'eccezionalità in quanto, come nella stragrande maggioranza dei Paesi europei, molti servizi e sistemi infrastrutturali sono stati realizzati per iniziativa e con fondi della collettività, allo scopo di dotare il nostro Paese delle necessarie condizioni per offrire a tutti i cittadini l'opportunità di beneficiarne. Accanto a ciò, si è tenuto conto, nel corso degli anni, dell'opportunità di sostenere alcuni settori produttivi considerati importanti e strategici. Del resto, il nostro Paese detiene queste partecipazioni senza infrangere alcuna disposizione comunitaria, in condizione di parità con gli altri *partner* europei. Il quadro normativo riguardante le società a partecipazione pubblica è complesso a causa dei diversi profili che intercorrono. Alla normativa societaria si sovrappongono gli effetti indiretti delle norme sul Patto di stabilità e la *spending review*, che condizionano gli enti pubblici che partecipano ai capitali delle società. Inoltre, incidono alcune normative di settore, principalmente di derivazione comunitaria, riguardanti la concorrenza e la liberalizzazione di taluni servizi. Occorre riconoscere che negli ultimi anni tutte le società in generale, e quelle partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici in particolare, hanno fatto doverosi passi nel segno della maggiore trasparenza, anche utilizzando le opportunità di maggiore fruibilità dei dati permesse dai portali Internet.

Su questo tema le aziende, soprattutto quelle che operano sui mercati competitivi, hanno fatto anche di più di quanto previsto dalla legge, per il motivo molto semplice che ciò permette, nei confronti dei *partner*, degli investitori, e degli stessi *competitor*, di presentarsi più forti e credibili rispetto ai mercati nei quali operano. I poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico e degli amministratori delle società partecipate sono disciplinate a livello generale dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale, (articolo 2449 del codice civile) prevede che se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Essa prevede inoltre che gli amministratori, i sindaci, o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono inoltre essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano poi in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista infine la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali, o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti. Alcuni importanti accorgimenti sono stati adottati dal legislatore per garantire che le società pubbliche siano orientate a criteri di efficienza, penalizzando gli amministratori che non agiscono con competenza e capacità; ne è esempio la previsione in base alla quale non può essere nominato amministratore di un ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006). Questo è quanto la legge è in grado di fare nel rispetto delle scelte di *management* che, se devono essere orientate dall'efficienza, devono tuttavia poter essere effettuate dagli amministratori che se ne assumono la responsabilità. Trovo pretestuoso che alcune mozioni presentate accusino lo Stato di poca trasparenza su questo tema. Sappiamo, infatti, che i principali dati relativi alle società a partecipazione pubblica sono disponibili e fruibili in diverse forme, compreso il canale Internet. L'elenco delle società per azioni partecipate da amministratori statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (all'appendice 4). Per quel che riguarda la parità di genere nelle società partecipate dallo Stato o da enti pubblici, la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e in particolare nei consigli di amministrazione delle società quotate in Borsa, dispone che le disposizioni dalla stessa previste si applicano anche alle società mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamento è quello adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251; ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti. In particolare, tale regolamento impone, come avviene per le società private e agli statuti delle società pubbliche non quotate, di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonei a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Veniamo infine ai criteri di reclutamento dei soggetti che dovranno rappresentare lo Stato negli enti partecipati; è chiaro che qui sta il nodo fondamentale. La competenza, l'indipendenza, la professionalità e l'integrità di queste persone devono essere assicurate con il massimo scrupolo, - permettetemi di dirlo - non credo che queste caratteristiche siano meglio garantite con le gare via *web* sul modello delle "quirinarie" tanto decantate da Grillo, che abbiamo poi scoperto essere un *flop* dal punto di vista della partecipazione, senza addentrarci nei retroscena e nei voltafaccia non appena i candidati si sono dimostrati non allineati al mentore. Già oggi, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi criteri e modalità rispettosi dei princìpi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Con gli impegni previsti dalla nostra mozione ci proponiamo di rafforzare i meccanismi di trasparenza e di selezione, senza scadere nel ridicolo o nel populismo. In particolare, proponiamo di impegnare il Governo: a disciplinare e a rendere pubblici - laddove non abbia già provveduto in tal senso anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo; ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari; infine, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rendere consultabili i *curricula* dei singoli candidati, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati. Mi sembrano tutte proposte di assoluto buonsenso, in sostanziale continuità con iniziative già avviate in tal senso dai precedenti Governi e assolutamente opportune e condivisibili.

lo sono per diversi motivi al centro del dibattito politico e che i nostri concittadini hanno ben presenti, rispetto ai quali chiedono a noi atti di coerenza e di coraggio. In particolare, queste mozioni investono il delicato rapporto tra la politica e l'economia, investono le forme con le quali lo Stato intende agire all'interno di questa attraverso le tante imprese che nel tempo sono state da esso promosse, nello specifico

che lo Stato deve esercitare, nel pieno delle sue funzioni, in vista del bene comune. Oltre a questo, le mozioni riguardano il tema della trasparenza, della competenza degli amministratori del rispetto della rappresentanza di genere: tante questioni cruciali - lo sappiamo bene - nel dibattito, ma anche per lo sviluppo del nostro Paese, per uscire da una situazione critica che non è soltanto di crisi economica, ma di crisi sociale e morale del Paese. L'economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente significative rispetto al quadro internazionale, di società partecipate, frutto di un'evoluzione storica improntata alla gestione di alcuni servizi e al sostegno di alcuni settori produttivi considerati strategici, non solo ai fini economici, ma anche per garantire dei servizi essenziali a tutti i cittadini. A ciò corrisponde un quadro normativo assai eterogeneo: al regime generale definito dal codice civile si sovrappone una serie di disposizioni di carattere speciale, introdotte attraverso interventi legislativi susseguitisi nel tempo. In materia di nomine nelle società partecipate è auspicabile, quindi, ed è il motivo del dibattito odierno, che si perseguano criteri di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità, attraverso il vaglio dei *curricula* e la loro pubblicazione, ai fini dell'esercizio di un controllo da parte del Parlamento e di tutti i cittadini, e la scelta di personalità competenti che non versino in situazioni di conflitto di interesse, allo scopo di scongiurare il rischio di pericolose commistioni tra politica ed economia, che pregiudichino il perseguimento del supremo interesse pubblico. È importante, cari colleghi, dare un segnale al Paese al fine di promuoverne la competitività, mettendo in primo piano l'esigenza di trasparenza nei procedimenti di nomina, premiando il merito nella selezione dei candidati, vietando il cumulo di incarichi, ponendo un tetto agli stipendi e soprattutto, nei casi di conferma, subordinando la nomina alla valutazione dei risultati. In questi ultimi anni, attraverso diversi interventi di carattere normativo, sono state introdotte (mi riferisco alle società non quotate e controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze) misure finalizzate al perseguimento di obiettivi di economicità della gestione, nonché di correttezza, trasparenza e funzionalità degli organi societari. novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società non quotate controllate dalla pubblica amministrazione, ha previsto che almeno un terzo dei membri di ciascun organo sociale appartenga al al genere meno rappresentato, stabilendo che per il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del regolamento tale soglia sia almeno pari ad un quinto; tratta di un'importante premessa per scardinare una tendenza molto diffusa, una situazione che si verifica nonostante l'eccellenza nelle donne sia ampiamente dimostrata. Infatti, ancora solo una donna compare alla presidenza tra le principali società partecipate del MEF che fanno capo allo Stato centrale; nessun amministratore delegato donna negli organismi partecipati da enti pubblici non economici, Ministeri e Regioni a statuto speciale. Nelle amministrazioni che detengono partecipazioni in consorzi o società la presenza femminile è davvero contenuta: soltanto il 13 per cento dei consiglieri. Non vi sono donne tra i presidenti degli organismi partecipati da agenzie fiscali, Monopoli di Stato, enti ex articolo

nei rimanenti organismi partecipati la presenza femminile nella carica di presidente varia da un minimo del 4 per cento ad un massimo del 7 per cento. Nessun amministratore delegato donna figura ancora negli organismi partecipati da istituzioni ed enti di ricerca, dai Ministeri, da Province e università, mentre nei restanti organismi partecipati le donne amministratore delegato sono tra l'8 e il 10 per cento. Voglio inoltre ricordare che, in attuazione della delega contenuta nella cosiddetta legge anticorruzione approvata dal Governo Monti (legge n. 190 del 2012), è stato emanato il decreto legislativo n. 39 del 2013, che interviene in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Tuttavia, il processo di riforma avviato, di cui ho citato le tappe importanti, deve indubbiamente essere completato attraverso misure che premino la trasparenza e la qualità delle modalità di indicazione dei componenti degli organi di amministrazione sotto il profilo della onorabilità, ai fini di assicurare la tutela dell'interesse pubblico, la corretta gestione delle risorse, la difesa dell'immagine del Paese. Il grado di discrezionalità nell'ambito della designazione dei componenti deve essere riequilibrato attraverso procedure atte a garantire che la selezione sia guidata da criteri assolutamente meritocratici attinenti le capacità e le esperienze professionali, escludendo così condizionamenti di sorta, men che meno di Se le politiche anticorruzione, in questo come in altri settori, avessero successo, assisteremmo alla crescita della fiducia dei cittadini tra loro e verso l'amministrazione pubblica. Aumenterebbe la nei confronti delle istituzioni circa la possibilità di contare sui propri meriti, cosa che in un periodo di crisi come questo è particolarmente rilevante. Per fare ciò concordiamo sul fatto che siano necessari i rigorosi siano necessari i rigorosi requisiti di onorabilità già previsti e l'introduzione di una specifica causa di ineleggibilità o di decadenza automatica in corso di mandato che escluda la presenza dagli organi di amministrazione di componenti nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio per talune gravi fattispecie di rilevanza penale, quali, ad esempio, reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica in materia tributaria e fallimentare. restano ferme le limitazioni già stabilite a legislazione vigente, come l'esclusione della nomina in quanto componenti degli organismi di amministrazione, di soggetti che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del consiglio di una Regione o di una Provincia autonoma o anche di enti locali con più di 15.000 abitanti. Al processo di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica deve corrispondere un processo di moralizzazione che riguardi tali società. È valutazione condivisa che la vigente disciplina delle società a partecipazione pubblica sia inadeguata, ma langue una seria discussione per l'auspicabile, generale riordino della materia; tra le tra le molte questioni, il disordine regolamentare, il prevalente approccio unitario ad una categoria di soggetti giuridici che omogenea non è, la mancata delle più innovative riforme tentate, una giurisprudenza

Ministro dovrebbe ascoltare gli interventi della discussione.Ce

con esportazioni che valgono la metà di quelle tedesche. Fondamentalmente ci sono quattro pilastri sui quali il nostro Paese vive come sistema industriale: le piccole e medie imprese (4,5 milioni di imprese che conosciamo); le grandi imprese industriali, delle quali giustamente la mozione di maggioranza ricorda anche i campi di attività (ben 32 società, che sono partecipate dal Tesoro, operanti

ma soprattutto le grandi imprese intervengono; quindi, il campo dell'energia, nel quale sono ancora presenti grandi imprese partecipate dallo Stato. Stato. Se c'è un problema che è sempre esistito è che questo sistema industriale non è mai riuscito a rappresentarsi nella sua integrità e interezza, sia in campo nazionale sia in ambito internazionale, a livello europeo come a livello extraeuropeo. Al Governo, però, viene sempre richiesto di fare strategie industriali per lo sviluppo, per la crescita, e facciamo le legislazioni in questa direzione.

Ora, se 32 sono le grandi aziende partecipate dallo Stato e operano nei settori che ho appena descritto, è immaginabile pensare che queste aziende siano nella linea delle indicazioni che il Governo e il Parlamento danno in termini di strategie industriali e che gli uomini che conducono queste aziende

Quello che mi preoccupa è che al riguardo nella mozione di maggioranza c'è scritto che il Ministro dell'economia dà conseguenti indicazioni impartite ai rappresentanti del Ministero nelle assemblee, che si configurano quali atti di alta amministrazione: il che vuol dire che i dirigenti indicati dal Ministero dell'economia danno alle loro aziende (che rappresentano, che conducono, che gestiscono e che guidano) indicazioni che provengono dal Ministero dell'economia. Io non sono sicuro che questo sia sempre accaduto; sia sempre accaduto; anzi, lo dico al neo vice ministro Fassina, ci siamo costantemente scontrati con un'inerzia burocratica che è appartenuta fino in fondo a quel Ministero, e che spesso non ci ha consentito di definire questi temi.

Noi non facciamo strategia industriale? La buona politica che riteniamo di rappresentare non fa strategie? Io voglio che vi siano condizionamenti della buona politica sulle grandi aziende di questo Paese e pretendo che i dirigenti indicati dal Ministero dell'economia in queste aziende rappresentino la buona politica e i condizionamenti che la buona politica è in grado di dare. Siamo solo cattiva politica? Non lo so.

accettiamola questa mozione. Spero sia animata da buoni propositi e che gli esiti siano largamente positivi, ma ricordiamoci lo dico perché rimanga agli atti qui per definire le strategie industriali di un Paese, che il Governo - qui rappresentato - le definisce e che gli uomini che saranno indicati dovranno essere all'interno di queste strategie. Questa è la priorità, al di là delle chiacchiere che si possono fare sul tema.

*(M5S)*. Presidente, vorrei portare l'attenzione dell'Assemblea su un aspetto specifico della mozione del Movimento 5 Stelle, cioè il passaggio in cui si fa riferimento alla legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. Questa legge, voluta da forze politiche diverse e giunta al traguardo dopo anni di intense battaglie che hanno riguardato e riguardano tuttora anche il *gender pay gap,* si caratterizza per due elementi: prevede una precisa gradualità di azioni e si pone un termine di dieci anni per raggiungere il suo obiettivo, la presenza di quote di genere negli organi sociali. Se ci interroghiamo sulle ragioni della gradualità e della durata predefinita degli effetti della legge n. 120, ci rendiamo conto che il legislatore non ha voluto configurare il provvedimento come la protezione di un genere (nella fattispecie quello femminile), cosa che in genere fa arricciare il naso a quanti, uomini o donne, sono convinti che il merito possa autogiustificarsi, autoregolarsi e, quindi, promuoversi da solo. Ha voluto, piuttosto, sostenere un processo tecnico riferito alla specifica realtà societaria, ma ancor più vuole essere culturale. Si considera che la legge, agendo nell'arco di tre mandati consecutivi, possa portare la presenza del genere meno rappresentato (quello femminile) dapprima ad un quinto, poi ad un terzo della rappresentanza degli organi societari, ottenendo un importante risultato culturale che si può e si deve misurare in termini di rinnovamento, maggiore meritocrazia e, dunque, più opportunità di crescita e sviluppo. Siamo convinti, infatti, che la presenza femminile possa portare un grande contributo al cambiamento di cui la nostra economia ha bisogno ora più che mai. Di cambiamento si tratta sia perché per recepire il contenuto della legge le società hanno dovuto provvedere a modificare i loro statuti (e questo non è solo un atto formale, ma implica un ripensamento della *governance*), sia per il valore numerico che queste modifiche impongono. In una realtà asfittica che negli anni ha visto una sorta di gioco dei quattro cantoni dei soliti personaggi passati da una società all'altra, entro l'arco di efficacia della legge dovrebbero entrare con ruoli chiave nelle società pubbliche circa 10.000 donne che avranno il compito di dimostrare di essere capaci di assumersi questa responsabilità. I principali detrattori della norma si sono trincerati dietro la presunta indisponibilità delle donne a ricoprire tali incarichi. Eccezione infondata, come dimostrano le raccolte di *curricula* di donne con elevati profili effettuate da svariate organizzazioni, ad esempio Ready for Board Women e tante altre, anche a livello locale. E qui veniamo a un altro aspetto che ci preme sottolineare: quello della selezione e dunque della possibilità di istituire nuove prassi e di introdurre nuovi criteri di scelta. Anche a livello societario, regole e criteri innovativi potrebbero avere una ricaduta importante sulle modalità di selezione del genere maggioritario, che oggi resta quello maschile. Trasparenza, merito, verifica delle competenze sono tutti termini che rimandano un'immagine agognata di efficienza e dinamismo. A questo fine associazioni autorevoli come la Fondazione Bellisario o istituzioni come il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno costituito banche dati di *curricula* meritevoli. stato virtuosamente recepito anche in realtà più piccole: ad esempio, a Reggio Emilia il dibattito sul tema è stato avviato per tempo, in collaborazione con il Comune, la Provincia e la Regione, e ha portato a un avviso pubblico per la presentazione di *curricula* di donne competenti, disponibili ad essere nominate nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali. La mozione del Movimento 5 Stelle nasce dalla contingenza del rinnovo del consiglio d'amministrazione di Finmeccanica, il cui rinvio consente al Senato di discutere il tema in tempo utile, ma ha comunque un più ampio e incisivo significato, alla luce del profilarsi dei rinnovi di organi amministrativi e di controllo in diverse società a partecipazione pubblica. Il processo virtuoso delineato dalla mozione, infatti, si applica anche alle altre società partecipate o controllate, che a breve vedranno un cambio nei consigli di amministrazione e di sorveglianza e nei collegi sindacali, ENI, ENEL, Poste Italiane e Ferrovie dello Stato, che sono centri di grande potere, ma anche - non dimentichiamolo - aziende pubbliche, che soprattutto in una situazione di ristagno economico potrebbero costituire un volano per l'intera economia italiana. Ciò che chiediamo sono candidature trasparenti, criteri resi pubblici, *curricula* disponibili e aperti al confronto e alla critica, assenza di conflitto di interessi e di opacità procedurali nella selezione e, infine, *curricula* di persone capaci Non abbiamo accolto con favore la notizia riportata informalmente dai giornali sulla possibilità che il Governo nomini un ennesimo comitato di saggi, come se il nostro Esecutivo avesse bisogno di badanti che legittimino le sue scelte. Si noti, a margine, l'inopportunità che un soggetto si scelga da solo chi deve dettargli i criteri a cui conformarsi. Piuttosto chiediamo che il Governo adotti come interlocutori, per la definizione dei criteri, i soggetti deputati a colloquiare con lui, parlamentari permanenti competenti per materia, cosa di cui non ci stancheremo mai di ribadire la necessità. Infatti è il Parlamento che ha la capacità di rappresentare i cittadini tutti e deve riappropriarsi di tale prerogativa, anche e soprattutto nelle fasi di nomina degli amministratori della *res publica* e nel controllo dei loro risultati. Permettetemi a questo punto di tornare su un punto centrale della nostra mozione: la promozione della presenza femminile in posizioni di rilievo e di responsabilità. È noto che le donne hanno minore mortalità scolastica e migliori risultati nello studio, ma è altrettanto noto che il genere femminile è di gran lunga penalizzato nel mondo del lavoro e delle professioni. Sono note, documentate e consolidate le statistiche che mostrano che l'Italia è fanalino di coda tra i Paesi europei, in relazione sia ai ruoli sia ai riconoscimenti tributati alle donne dal cosiddetto mondo produttivo. Concludo con un'ultima considerazione: voglio ricordare che oggi abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul, che si occupa di un'emergenza, quella della violenza contro le donne, e giustamente è stato richiamato il fatto che il rispetto della donna si costruisce, prima ancora che nell'emergenza, con un approccio culturale profondo. La legge n. 120 del 2011 ci mette di fronte alla responsabilità di accreditare le donne anche nell'eccellenza, per dare luogo a un cambiamento culturale profondo, che restituisca non solo dignità piena nella realizzazione professionale e retributiva,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, condivido anch'io lo spirito del senatore Romani nella lettura

forme indebite di pressione che rendano più difficile l'individuazione e poi la designazione di personalità adeguate per la guida delle grandi imprese nelle quali lo Stato esercita il controllo, di diritto o di fatto, in forma singola ovvero in forma congiunta quando aderisca a patti con altri azionisti. Ma tant'è: a questo punto ritengo inutile fare i processi alla buona e alla cattiva politica. ha la sua storia, è in questa storia c'è stato, per esempio, il caso dell'amministratore di una grande azienda pubblica che finì la sua vita emarginato da tutto per un processo di Tangentopoli, colui il quale aveva organizzato il pagamento della mazzetta è poi diventato l'amministratore della società che era stata corrotta. La nostra, quindi, non è una storia perfetta e di uno scudo c'è bisogno: la domanda è se questo scudo è organizzato nel migliore dei modi o se possa essere ulteriormente perfezionabile.

Il primo fa riferimento ai requisiti di onorabilità che vengono giustamente richiamati e posti in evidenza. Credo che la parte che riguarda i vincoli alla scelta dei nuovi membri dei consigli di amministrazione indicati dal Ministero dell'economia vada bene. Penso invece che, là dove si prevede la decadenza automatica in corso di mandato, vada meglio definita la posizione, ovvero non credo che una condanna penale, di cui non si specificano l'importanza e la consistenza, basti di per sé a determinare la decadenza. Ritengo più corretto adottare, a questo proposito, la normativa da tempo in vigore nel settore bancario, che poi è stata estesa a quello assicurativo. Faccio presente che banche e assicurazioni trattano la materia più delicata oggi presente nell'economia, ossia il risparmio, che è costituzionalmente garantito. Credo sia corretto prevedere la sospensione in automatico dell'amministratore condannato per quei reati di cui abbiamo detto

se lo crede, nel caso in cui il consiglio di amministrazione e l'assemblea stessa si assumano la responsabilità di decidere che questo è bene per la società.

La storia delle aziende pubbliche è stata costellata di diarchie disastrose, nelle quali presidenti con pieni poteri facevano la guerra ad amministratori delegati con pieni poteri o nelle quali presidenti di campanello dovevano dirimere eterne liti fra due o tre amministratori delegati. Credo che queste storie non si debbano ripetere. Invito, pertanto, ad estendere

distinzione dei ruoli e la specificazione delle competenze proporrei ai colleghi, che hanno steso con meritorio impegno e tanta fatica

l'impegno che gli amministratori dal Ministero stesso designati promuovano un'analoga attribuzione delle deleghe nel rispetto dei diritti dei soci

una trasparente, ottimale ed equilibrata organizzazione delle società a partecipazione pubblica che costituiscono nella realtà economica del nostro Paese un rilevante punto di riferimento. Dette società, infatti, rappresentano per lo più realtà industriali di grande peso che ci rendono competitivi e, in alcuni casi, sono anche *leader* a livello mondiale (mi riferisco a ENEL, ENI, Finmeccanica); inoltre, a livello occupazionale sono una realtà certa e consolidata. In Italia, ben 32 società sono partecipate o controllate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre altre sono partecipate o controllate da Regioni ed enti locali. Per ciò che riguarda l'elezione dei membri del consiglio chiediamo al Governo di stabilire criteri e modalità per le nomine e la decadenza dei componenti dei consigli di amministrazione che tengano conto

condanna per reati contro la pubblica amministrazione) e la decadenza automatica durante il mandato di coloro che abbiano ricevuto una condanna penale o che abbiano patteggiato la pena per quel reato di amministrazione di membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del consiglio regionale, di una Provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazioni superiori ai 15.000 abitanti. Per quanto riguarda la valutazione dei requisiti professionali, si richiede un *curriculum* con esperienze analoghe al nuovo incarico nel consiglio di amministrazione e nessun conflitto di interesse o cumulo di cariche in società concorrenti. inoltre una nutrita serie di requisiti al fine di contribuire nel massimo della trasparenza ed efficienza all'ottimo assetto del Un altro impegno che chiediamo al Governo è di riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in merito al rispetto dei criteri segnalati nella mozione. Ebbene, alla luce di quanto esposto, darò il mio voto favorevole, augurandomi il consenso di tutti i colleghi, perché ci tengo a ribadire che questa mozione si muove nella direzione della correttezza,

onorevoli senatori, sono d'accordo anch'io che questa mozione, che ha il pregio di sintetizzare e di enunciare principi molto importanti in materia di nomina nelle società pubbliche, riguardi un aspetto non decisivo del sistema delle società partecipate. Sono d'accordo che il tema vero e più grande sia quello delle società pubbliche. È la storia dell'intervento dello Stato nell'economia, una storia con luci e ombre, ma una storia che ha avuto un suo inizio con l'IRI, un suo sviluppo attraverso la privatizzazione degli anni '90 e doveva avere un suo sviluppo anche con le liberalizzazioni. Un processo che è stato fermato; fermato; uno stop ad un processo che doveva modificare la presenza dello Stato in questi settori. Questo non è avvenuto per responsabilità degli articoli 41 e 43 della Costituzione che, in realtà, hanno consentito l'intervento dello Stato nell'economia, che è stato per molti versi risolutivo. Ma il tema delle società pubbliche è davvero un tema su cui fare una riflessione profonda non solo focalizzando l'attenzione sulle società statali, ma anche sul tema delle società partecipate dei Comuni. Dimenticare che c'è una riflessione che riguarda anche questo tipo di intervento pubblico nell'economia sarebbe assolutamente miope. Siamo di fronte, in questo ambito, ad un sistema che ha creato danni enormi. Ricordo "per cittadinanza" il caso delle società partecipate del Comune di Parma, ma so che non è l'unico caso. Voglio ricordare che, al di là e oltre il tema del "buco" nelle casse pubbliche, questi fenomeni incidono anche sui diritti dei cittadini perché stanno portando i Comuni a chiudere servizi, scuole

che rispetto all'intervento pubblico nell'economia facessimo una riflessione più ampia, semmai la dovessimo avviare, perché c'è un tema di privatizzazione delle funzioni pubbliche, un tema sul piano della Costituzione materiale di riflessione sui ruoli

bancarie che ci conduce alla necessità di una riflessione organica sull'intervento dello Stato nell'economia, a una riflessione su un sistema che non si ferma ai requisiti delle nomine, che è più ampia. Mi auguro che questo sia un tema che venga affrontato. Il tema dei requisiti per le nomine è in questo quadro e allo stato dell'arte importante, ma non deve distrarre dalla necessità di una riforma complessiva del sistema dell'intervento pubblico nell'economia. Le ragioni ci sono tutte perché sono molti i fenomeni distorsivi e le forme di ricorso alla società per eludere principi e responsabilità proprie dell'enti pubblici, per sviluppare E credo che sotto questo profilo si debba denunciare anche con molta chiarezza che le distorsioni denunciate anche in questo dibattito nel rapporto tra Governo e amministratori nominati dal Governo anche un tema del modo in cui queste relazioni sono state approcciate e anche una questione relativa al modo in cui si è preteso

degli amministratori delle società, esempi negativi e, nell'ambito dei comportamenti degli uomini di Governo, troppo spesso la pretesa di prevaricare e di non avere avere professionisti alla guida di dette società, ma degli "*yes* *men*". Di questo l'Italia non ha bisogno. Di questo il sistema economico italiano non ha bisogno. L'augurio è che, passando per questa importante per questa importante mozione, si arrivi ad una riflessione più ampia, ad una riflessione che ci possa portare a ridisegnare davvero l'intervento dello Stato nell'economia.

i cui testi sono stati già stampati e sono in distribuzione. Ha facoltà di parlare il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Fassina, al quale chiedo di esprimere il

consente di fare un importante passo in avanti. Negli ultimi anni sono stati approvati provvedimenti che hanno consentito un miglioramento nelle procedure di nomina e nelle scelte, ma certamente le mozioni

il punto 2, che chiede la pubblicazione sul sito del Ministero di tutti i *curricula* pervenuti, rischia di limitare la possibilità di di candidature, data la sensibilità di queste scelte rispetto alle posizioni occupate da coloro che si si presentano per concorrere alla nomina in una società pubblica. Per quanto riguarda poi il punto 3, riteniamo che si possa correre il rischio di scaricare sulle procedure di nomina una eccessiva tensione politica, che potrebbe andare a scapito della qualità delle scelte che vengono fatte. parere negativo anche sulla mozione di cui è primo firmatario il senatore Bitonci, in particolare per quanto riguarda l'impegno previsto per il Governo al punto 2, per le ragioni che ho appena richiamato, essendo tale punto

Esprimiamo invece parere favorevole sulla mozione di cui è primo firmatario è il senatore Tomaselli. mi pare recuperi i punti importanti delle mozioni precedenti, evitando, al tempo stesso, quegli elementi di rigidità che ricordavo prima. Essa indica dei criteri che possono portare alla massima trasparenza e ad un miglioramento rilevante, come ricordavo all'inizio, delle procedure di selezione delle persone, dei consiglieri di amministrazione e dei presidenti (quindi, auspicabilmente, anche ad un miglioramento delle *performance* aziendali). Rispetto ai punti che sono stati sollevati nel corso della discussione, credo ci siano osservazioni importanti che vanno tenute in considerazione. alle riflessioni del senatore Romani rispetto alle strategie industriali e al dovere della politica - della buona politica - farsi carico delle strategie industriali. Anzi, credo che se c'è stato un *deficit*, negli anni che abbiamo alle spalle, nella possibilità di indicare strategie industriali, è una funzione che la politica deve riconquistare, nel rispetto - ovviamente - del suo ruolo, cioè, appunto, quello di indicare strategie e non di fare le scelte specifiche del giorno per giorno.

non è mai pervenuto.

credo che questo sforzo vada fortemente sostenuto e anche apprezzato da parte di tutti e - spero - anche dell'opinione pubblica, perché vogliamo dare al Paese un segnale di unità di tutte le forze politiche quando si tratta di dettare le regole di comportamento della politica nelle scelte di alta amministrazione del Paese. Quindi condivido e mi auguro - anzi, sono fiducioso - che si possa arrivare a questo auspicato testo 4 nei tempi consentiti, che la Presidenza valuterà.

quali verificheremo il ritiro degli emendamenti conseguenti a questo testo unitario. Quindi, chiederò il parere del Governo.

Presidente, ci troviamo oggi di fronte a un atto molto importante nel rapporto Governo-Parlamento, ed è un decisivo passo in avanti per la trasparenza. *(Brusìo)*. Ma la pregherei, Presidente, visto che c'è poco tempo, di invitare

e nella trasparenza delle modalità di adozione delle decisioni del Governo in materia sia di nomine sia di *governance* delle società pubbliche. Di questo va dato atto al ministro Saccomanni e al vice ministro Fassina, che ha interloquito con grande attenzione

e che, proprio per questo, devono essere gestite con criteri manageriali, senza cedimenti a interessi di parte o a logiche opache e clientelari. Si tratta di settori molto diversificati (industriali, di servizio, di gestione di attività pubbliche) le privatizzazioni nel corso degli anni hanno ridotto il perimetro dello Stato imprenditore, ma ciò nonostante le società partecipate di primo e secondo livello rimangono ancora molto, molto estese. È un perimetro amplissimo e su alcune è intervenuta la *spending review* con modifiche molto incisive, quanto ad ampiezza dei consigli di amministrazione, un tempo dilatati a dismisura, di composizione, ormai riservata solo ai funzionari dello Stato, di livello dei compensi e di presenza delle donne. Ma non ci si può nascondere che accanto a queste realtà di eccellenza, molti di questi organismi societari sono serviti, negli anni, ad aggirare le regole pubblicistiche in materia di appalti e di assunzioni, ad occultare il debito, a gestire in modo talvolta clientelare settori rilevanti dell'attività pubblica e delle relazioni con il mercato e con gli interessi economici. Oggi le mozioni che noi stiamo per votare tentano di vincolare l'azionista pubblico rispetto a criteri severi di professionalità e di onorabilità, che in parte erano stati anticipati nella direttiva Grilli. È un passo importante. Siamo certi che il Ministro vi si atterrà, ma spetterà al Parlamento attrezzarsi per vigilare che questi criteri siano effettivamente rispettati in tutta non possiamo nasconderci che il sistema delle società pubbliche è percepito dall'opinione pubblica come parte di quella casta i cui privilegi hanno separato le istituzioni e la politica dall'opinione pubblica,

Per questo oggi noi riteniamo necessario dare un segno netto e deciso di discontinuità e di resipiscenza della politica nel segno della moralizzazione, della separazione della politica dall'economia, della abolizione del principio di inamovibilità e, al contempo, anzi, direi proprio per questo, della valorizzazione del grande patrimonio imprenditoriale, manageriale, professionale e tecnologico custodito in molte di queste società. Per questo la valutazione finale di Scelta Civica dipenderà dall'accoglimento o meno dei due emendamenti che, a nostro avviso, condizionano questo elemento di discontinuità. Quello che impedisce agli ex parlamentari o ex eletti di essere travasati automaticamente nei consigli di amministrazione e quello che limita il principio di inamovibilità e quindi la permanenza nello stesso incarico a tre mandati, cioè a circa un decennio, salvo ovviamente che il Ministro ritenga Grazie

Presidente, anche noi attendiamo di conoscere l'opinione del Governo sul testo che è in fase di

perché, pur condividendo la gran parte dei contenuti che sono presenti, anche se in modo differente, in tutte le mozioni che sono state presentate, a noi pare - e lo diciamo al Vice Ministro, in particolare - che ci sia un problema di semplificazione reale sia del sistema delle partecipate e delle controllate sia degli organi di governo di questi soggetti. Dovremmo andare sempre di più verso l'individuazione di organi monocratici, competenti sul piano professionale, che garantiscano i risultati che il Governo, nazionale, regionale, locale, attribuisce come obiettivi a quei soggetti, e che, nella gran parte dei casi, possa assolvere insieme alle funzioni di amministrazione generale come a quelle di direzione generale delle strutture. Riteniamo che questo sia il vero segnale che ci si deve attendere anche da una coalizione come la vostra,

minoranza; adesso ci sono sempre due relatori di maggioranza. Se il criterio è che l'amministrazione si adegua alle esigenze di funzionamento politico delle coalizioni e questo sistema noi lo ripetiamo dalle Aule del Parlamento fino agli organi esecutivi e finanche nei consigli di amministrazione dei gestori finali, cioè nel sistema delle partecipate e delle controllate, siamo alla rovina: altro che semplificazione, faremo un prodotto di complicazione aggiuntiva a quella che già subiamo, e non è la strada giusta per risolvere i problemi. Problemi che rimangono - lo dico

a livello locale, hanno problemi di sopravvivenza, che sono dettati dalla legge, ma hanno anche problemi di occupazione, perché molti di coloro che operano soprattutto nelle società *in house* nelle società *in house* provengono dai bacini dei lavoratori socialmente utili, che sono stati recuperati, attraverso quel sistema, all'occupazione. Ebbene, noi rischiamo di trovarli di nuovo per strada ad incrementare quel numero ormai enorme

Signor Presidente, la questione delle società partecipate nel nostro Paese è un po' il frutto tutto italiano dell'evoluzione storica, storica, a sostegno di alcuni settori produttivi che allora si giudicarono strategici. Partiamo dal salvataggio delle due banche: la Banca commerciale italiana, il Credito italiano; nel 1926 viene fondata l'AGIP per assicurare autonomia nel campo energetico; nel 1933 l'Istituto per la ricostruzione industriale; nel 1950 la Cassa per il Mezzogiorno; l'ENI nel 1953, per arrivare nel 1956 addirittura ad istituire il Ministero delle partecipazioni Cosa ha significato? Una grossa ingerenza dello Stato nell'economia e, chiaramente per l'azionista pubblico, i poteri di nomina, disciplinati poi dalla dalla codicistica civile, cioè viene attribuita la facoltà di nominare amministratori, nonché sindaci, in numero proporzionale alla partecipazione.

Grazie

un amministratore privato se lavora male fallisce, mentre il fallimento per gli amministratori pubblici

Oggi discutiamo e ci concentriamo particolarmente sulla conseguenza della legge n. 120 del 2011, cioè sulla scarsa presenza all'interno delle società pubbliche delle donne. La minestra è stata qui allungata con

garanzia di applicazione sarebbe stata innanzitutto l'informazione e la conoscibilità. E cosa stiamo portando a casa? Non molto, perché abbiamo dovuto convergere su un testo unificato, per cui non ci sarà più l'obbligo, per esempio, della

care colleghe, cari colleghi, è innegabile che stiamo vivendo un periodo di transizione per la politica, in cui vecchie logiche sono state rimesse in discussione, potremmo quasi dire «a furor di popolo». Il Movimento 5 Stelle e i suoi 8 milioni e mezzo di elettori sono la diretta conseguenza della necessità condivisa di portare avanti un processo di profondo rinnovamento, che vuole riportare gli interessi del cittadino al centro del dibattito politico. Chi non è sordo alle piazze, chi è continuamente e strettamente a contatto con i cittadini, non può certamente non accogliere le istanze che emergono a gran forza dai nostri elettori: onestà, legalità, trasparenza, meritocrazia devono ora entrare prepotentemente nella gestione della cosa pubblica. Il Movimento 5 Stelle ha fatto di questi valori la propria bandiera e, paradossalmente, ben prima che noi entrassimo in Parlamento gli altri partiti si sono fatti promotori di tardivi e incompleti richiami, ad esempio, alla questione morale, al contenimento dei costi della politica e a processi di selezione meritocratici. Se hanno fatto questo, ciò questo, ciò è anche merito nostro. A proposito di meritocrazia, affrontiamo dunque il grande tema delle nomine dei vertici delle società a partecipazione statale, oggetto delle mozioni che stiamo dibattendo in quest'Aula. I recenti scandali giudiziari che hanno coinvolto la società Finmeccanica hanno posto con forza il problema delle nomine dei vertici, fino adesso effettuate prestando poca attenzione a criteri come l'incompatibilità con incarichi politici, l'assenza di conflitti d'interessi, l'esperienza, la competenza e così via. relative a Finmeccanica, avvenute in piena campagna elettorale, hanno riproposto quindi con forza il tema dell'onestà dei cosiddetti *manager* e di chi li ha messi al loro posto: un problema enorme di mancanza di senso dello Stato, che si avvertiva. Il Governo attuale ha rinviato la nomina del nuovo presidente e, nel corso dell'assemblea di Finmeccanica di poche settime fa, è stata rimandata a luglio la nomina dei due consiglieri e sono stati fatti dei generici e blandi richiami alla trasparenza. Le buone dichiarazioni di intenti rischiavano di rimanere lettera morta e di produrre risultati insoddisfacenti se il Parlamento non fosse intervenuto a sedare il braccio di ferro, tutto politico, intorno ai tre quattro candidati, che era sotto gli occhi di tutti e che costituiva il reale motivo della decisione di non decidere assunta fino adesso. il Movimento 5 Stelle rivendica il merito di aver avviato il dibattito parlamentare sulle nomine: chissà quanto tempo sarebbe passato, se non fosse stato per noi.

domanda, e quello sulla turnazione del comitato di garanzia, per garantire che i membri di questo importante processo nell'opera di selezione cambino ogni tre anni. Tutti questi emendamenti sono stati accolti e per questo motivo abbiamo ritirato la nostra mozione, che è confluita in quella della maggioranza. Dunque oggi, cari colleghi e colleghe, in quest'Aula abbiamo finalmente la possibilità di realizzare un nuovo corso ‑ lo sottolineo: un nuovo corso ‑ nella scelta delle nomine dei vertici delle società partecipate dallo Stato, improntato finalmente a iriteri di trasparenza e meritocrazia, nonché alle pari opportunità di genere. Duole considerare che questa possibilità sia maturata solo a seguito di svariate inchieste giudiziarie e di cospicue perdite finanziare del gruppo Finmeccanica e di altri che non hanno mancato e non mancheranno di avere ripercussioni anche sul piano lavorativo per le migliaia di dipendenti del gruppo e per le loro famiglie, la cui responsabilità, ricordo, non può che ricadere interamente sulle spalle di chi ha avuto il compito di nominare prima e di controllare poi la dirigenza del Il Gruppo del Movimento 5 Stelle ‑ e concludo, signor Presidente - con il voto favorevole a questa mozione vuole essere portavoce di tutti quei cittadini che, vedendosi richiedere titoli su titoli, competenze su competenze, *curricula* su *curricula*, anche per fare i lavori più semplici, si sentono profondamente umiliati quando gli stessi criteri vengono completamente disattesi, qualora si tratti di assegnare, invece, incarichi ben più importanti, che hanno a che fare con la gestione dei pubblici interessi e del pubblico denaro. *(Vivi

Onorevoli colleghi senatori, come evidenziamo in questa mozione, le società a partecipazione pubblica rappresentano una risorsa per il Paese

e non deve rinunciare ad esercitare un'azione di supporto alla libera impresa, ma deve essere promotore di crescita e sviluppo socio-economico, attraverso le proprie iniziative volte a rafforzare il sistema Paese.

Lo Stato in particolare, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, detiene la partecipazione diretta di maggioranza o controllo di 32 società operanti in settori strategici,

l'ENI, la Cassa depositi e prestiti, le Ferrovie dello Stato e la Finmeccanica, società che rappresentano un'importante presidio di occupazione e assumono una posizione *leader* a livello mondiale. L'articolo 4, al comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dispone che nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo politico ed amministrativo gli organi di Governo provvedano in particolare ad effettuare le nomine, le designazioni e atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni. Per tali necessità è quindi opportuno che siano incrementate le disposizioni che possono garantire la trasparenza e la qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica e rafforzare i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori stessi, escludendo il rischio di indebita e nociva intromissione politica che possa compromettere l'esistenza e la natura societaria degli organismi controllati. È quindi necessario che il Ministro dell'economia e delle finanze per le società controllate direttamente o indirettamente dal medesimo Ministero possa fare fare affidamento su criteri e modalità di carattere generale per la nomina e la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione, in modo da assicurare anche il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, all'introduzione di una specifica causa di ineleggibilità per coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio o che abbiano patteggiato la pena o riportato una condanna per talune gravi fattispecie di reato, quali

dei componenti degli organi di amministrazione nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna penale o che abbiano patteggiato la pena per le suddette fattispecie di reato. Mi riferisco infine all'esclusione dalla nomina a componenti degli organi di amministrazione di membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una Regione e di una Provincia autonoma superiore a 15.000 abitanti. Tutto quanto sopra si basa anche sugli interventi legislativi più recenti, che hanno comportato una sottoposizione delle società pubbliche non solo a misure di contenimento della spesa, ma anche a regole di trasparenza e vincoli di organizzazione. Tale assetto normativo, venuto delineandosi nel tempo, non sembra tuttavia aver assunto fino ad oggi le caratteristiche di un sistema organico e stabile. Anche a fronte di tali ragioni, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo del PdL, nell'auspicio che si possa addivenire quanto prima ad una più completa definizione della

Signor Presidente, colleghi, questa è una mozione innovativa, perché individua requisiti di professionalità e onorabilità con vincoli stringenti, ma anche *governance* snelle, compensi ridotti degli organi amministrativi e un importante equilibrio di genere. A breve avremo 199 nomine, a cui si potranno applicare questi criteri. Partendo dall'amministratore delegato delle società,

troppo spesso avviene che, in entrata e uscita da società, si abbiano interessi omologhi o contrastanti. Abbiamo visto in passato che soggetti controllori sono diventati attori in società operative controllate in precedenza o, peggio ancora, abbiamo visto decisori pubblici prendere posizioni operative in società private. Credo che un periodo di decantazione sia necessario per il passaggio tra pubblico e privato e viceversa. Il presidente deve avere un adeguato equilibrio

voglio sottolineare, perché, se è vero che nel passato possono esserci stati eccessi, è anche vero che spesso alcune società si devono confrontare sui mercati mondiali, e la *governance* deve avere l'esperienza, la professionalità, la visione industriale, economica e finanziaria per competere sui mercati internazionali; quindi, le scelte devono tenere presenti questi parametri, che richiedono adeguate remunerazioni. Voglio ancora sottolineare l'importanza dell'istituzione di un comitato di garanzia che dovrà effettuare le scelte, composto anche in questo caso da personalità di riconosciuta capacità e competenza, dopo un'istruttoria approfondita. Credo sia molto importante - mi rivolgo al Governo ma anche a noi stessi - l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di analoghi criteri e procedure. In questo caso abbiamo visto troppo spesso nelle società controllate dagli enti e nelle municipalizzate nomine fatte con i soli criteri di appartenenza, in cui spesso i consigli di amministrazione sono un *refugium peccatorum* per i non eletti e gli amministratori rispondono all'azionista ente i non eletti e gli amministratori rispondono all'azionista ente con pratiche clientelari sia nelle assunzioni che nelle politiche economiche e industriali delle stesse.

Vorrei chiedere al Vice Ministro di dire due parole sul motivo del suo parere negativo

Che prima di ogni votazione ciascun senatore può fare un annuncio di voto. DELLA VEDOVA *(SCpI)*. Abbiamo stabilito i cinque minuti sulla dichiarazione di voto, ma non che non ci sarebbero state dichiarazioni di voto. PRESIDENTE. È stata accolta all'unanimità l'armonizzazione dei tempi, che prevede per le ore 19.30 il voto.

il voto favorevole sulla mozione all'approvazione di questi emendamenti per la ragione fondamentale - mi rivolgo ai colleghi e al vice ministro Fassina che se vogliamo fare un passo avanti, sapendo benissimo che non discutiamo di principi, ma stiamo a discutere in base a quello che realmente è successo in Italia nella gestione delle aziende pubbliche, dalle più grandi alle più piccole, perché non mettiamo, signor Vice Ministro, un diaframma di un solo anno tra gli incarichi parlamentari ed elettivi e la nomina nei consigli di amministrazione?

può essere catturato non solo dalla creazione di valore per le aziende, ma anche da tutte le altre pratiche che la realtà italiana consegna. Semplicemente non capiamo perché non inserire questi due elementi, formulati in modo ragionevole, in questa, per il resto, condivisibile mozione. Ma se non si ha il coraggio di fare questi due passi - lo dico al Vice Ministro - noi ci asterremo.

resto appare evidente, in considerazione anche della complessità dell'argomento e degli interventi ad esso integrati, in particolare modo in una situazione complessa per il Paese, nella quale i professionisti non mancano e si assiste ad un blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione,

porre a quest'Aula un problema che si porrà, da adesso in avanti, per una categoria non piccola di cittadini italiani. L'11 giugno il Parlamento europeo ha proceduto all'approvazione del regolamento n. 353, con il quale ha sostanzialmente declassato i celiaci e la loro malattia a una moda.

i prodotti destinati ad alcune categorie vulnerabili della popolazione, che comprendono i lattanti, i bambini, chi ha fini medici speciali, chi deve perdere peso, ma non ha contemplato i celiaci.

riferimento non sono supportate da concreti studi scientifici. Queste stime fanno riferimento, in particolar modo, a una percentuale non ben nota della popolazione che soffrirebbe soltanto di sensibilità

un ordine del giorno e che erano state presentate delle mozioni per chiedere al Governo un provvedimento urgente in materia di clausola di salvaguardia, per far in modo che la nostra agricoltura fosse salvaguardata dalla possibilità di

alla clausola di salvaguardia, questo non è accaduto. Sono state fatte interrogazioni urgenti, ma non è accaduto niente.

che molti di noi ben conoscono. È stato seminato mais OGM, quindi geneticamente modificato, con i grandi problemi che ciò potrà arrecare di nuovo alle produzioni nel Friuli. Vorrei infatti ricordare

e provvedere immediatamente ad approvare la clausola di salvaguardia.

e dei trasporti, il 23 maggio, su un'opera importante come l'Arcisate-Stabio, un'opera che sta incontrando dei problemi significativi. A tutt'oggi non è giunta alcuna risposta e alcun riscontro in merito. È naturale che quando un parlamentare presenta un atto di sindacato ispettivo significa che c'è un problema e che quest'ultimo deve essere preso sul serio, altrimenti vorrebbe dire derubricare la nostra stessa attività semplicemente a corollario rispetto a quella del Governo. Quindi l'invito naturalmente è quello, attraverso questo intervento e attraverso la sua la sua persona, a sensibilizzare il Governo affinché agli atti di sindacato dei parlamentari corrispondano delle risposte concrete ed esaustive. Siamo disposti anche ad accettarne altre forme rispetto a quella scritta, come può essere quella orale, ma certamente non siamo disposti ad accettare che ai cittadini vengano dati semplicemente dei tempi di attesa, senza che vi sia alcuna attività di governo e soprattutto senza che ci sia alcuna risposta.

determina che resta a verbale. Questo non modifica l'esito della votazione e il proprio voto favorevole o contrario non viene commutato rispetto agli stampati elettronici, che sono l'unico documento che resta.

rivolgendo alla nostra Regione. Quindi, nei giorni scorsi siamo rimasti veramente molto sorpresi che ancora adesso, giugno 2013, un Ministro dell'ambiente, peraltro giovane, dica che per risolvere il problema dei rifiuti in Campania e per non andare in procedura d'infrazione con l'Europa dovremo costruire ancora due inceneritori, quando l'Europa del Settimo programma non ci chiede inceneritori, perché non li prevede per il 2020: per quella data prevede il divieto di incenerire. Allora vorrei fargli arrivare questa notizia, perché probabilmente non è bene informato e mi dispiace: l'Europa ci chiede ben altro! Gli inceneritori sono fuori mercato e hanno un senso economico solo perché ancora hanno incentivi CIP6. Per inciso, la Campania, a detta dell'assessore all'ambiente Romano, è attualmente a un livello di raccolta differenziata che la colloca al quarto posto nel panorama nazionale. Delle due cose è vera solo una: o siamo in infrazione con l'Europa oppure siamo al quarto posto come raccolta differenziata. Vorrei un chiarimento, altrimenti mi confondo; ho bisogno di un po' di certezze. Quindi, cosa vogliamo fare? Vogliamo cominciare oggi a costruire macchine che producono danni ambientali incredibili, danni economici incredibili al territorio, danni alla salute? Cominciamo oggi a costruirli e li avremo tra sei anni: 2013 più sei quanto fa, Presidente? Mi dispiace, ho qualche difficoltà, forse perché sono influenzata, però mi sa che siamo vicino al 2020, quindi poi dovremo chiudere gli inceneritori. *(Applausi dal Gruppo zero rifiuti e zero combustione e, quindi, impianti di compostaggio. In Campania abbiamo bisogno di impianti di compostaggio. *(Applausi ministro Ronchi, ma nessuno è aperto. Siamo in questa situazione: non abbiamo impianti di compostaggio. Per questo l'Europa ci sanziona, perché portiamo ancora fuori i rifiuti a causa del fatto che non abbiamo impianti di compostaggio. Volevo fare arrivare questa notizia al Ministro.